L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta

Gentili senatrici e senatori, è con sentimento di sincero affetto e commozione che desidero ricordare in quest'Aula il professor Francesco Alberoni. Alberoni. Come sapete, egli era un sociologo, uno scrittore, un giornalista, un docente universitario. Francesco Alberoni è stato un protagonista veramente importante del panorama culturale della nostra epoca e soprattutto uno dei più intelligenti osservatori e acuti interpreti della nostra società. Nel corso della sua lunga carriera accademica, Francesco Alberoni ha ricoperto la cattedra di sociologia in alcune delle più importanti università italiane e internazionali, dalla Cattolica di Milano all'Università di Losanna, dall'Università di Catania alla Statale di Milano, diventando un irrinunciabile punto di riferimento per generazioni di studenti e anche di docenti. Verso la fine degli anni Sessanta ha ricoperto, con autorevolezza, il ruolo di rettore dell'Università di Trento, impegnandosi sia nel potenziarne il suo ruolo come istituto superiore di scienze sociali, sia nello sviluppo di un modello universitario più moderno e attento al coinvolgimento degli studenti nelle scelte didattiche. Dopo il suo ultimo incarico accademico come rettore dell'università IULM di Milano, che si concluse nel 2001, Francesco Alberoni ha continuato con passione e generosità il suo impegno culturale e scientifico nei consigli di amministrazione di Cinecittà e della Rai e, infine, come Presidente, per oltre dieci anni, dal 2002 al 2012, del Centro sperimentale di cinematografia. Uomo di grande saggezza e profonda empatia, con le sue opere Francesco Alberoni ha esplorato le sfumature più complesse delle relazioni umane. Le sue teorie, notissime, sull'amore, sull'amicizia, sulla società hanno affascinato e ispirato milioni di lettori in tutto il mondo. Un successo dovuto anche alla sua capacità di esprimere concetti complessi con parole semplici, comprensibili a tutti: una grande dote, che Alberoni aveva e che ci ha tramandato. Ho avuto il privilegio personale di conoscerlo, non soltanto nella fase degli ultimi anni della sua vita, quando aveva deciso di candidarsi politicamente a Milano e anche alle elezioni europee, non per essere eletto, ma per partecipare, anche se poi risultò eletto. Io l'ho conosciuto molti anni prima, quando era nel pieno della sua attività accademica, lui insieme alla sua compianta moglie, e ne ho tratto sempre un'impressione di grande forza, di grande intelligenza, ma soprattutto di grande umanità. Quello che lo ha contraddistinto, almeno nel rapporto personale che ho avuto con lui, è stata sempre questa grande umanità e l'importanza che dava a sentimenti come amicizia, fiducia e solidarietà, che in una comunità sono un elemento che dà forte coesione. Con Alberoni salutiamo un uomo che ha reso onore all'Italia e che, come hanno testimoniato le tante persone che hanno voluto rendergli un ultimo saluto in occasione dei suoi funerali a Milano, ha lasciato dietro di sé un'importante traccia di affetto, insieme ad un'eredità di idee e di valori che, sono certo, continuerà a ispirare anche le future generazioni. Concludo rinnovando il mio affetto, il mio cordoglio e la mia vicinanza

Nel commemorare una persona che si ammira tantissimo, che ha influenzato, con la sua immensa cultura, la mia piccola cultura

Mi sento in colpa per le poche cose che dirò, ma anche per le cose che non dirò. Descrivere infatti in pochi minuti, in questa Aula, una vita così importante ti fa sentire in qualche modo inadeguato. Io credo che Francesco Alberoni abbia tanti meriti; intanto quello di aver manifestato il suo disagio da studente. Non era d'accordo con le regole imposte, voleva una scuola più liberatoria, più all'altezza del piccolo bambino e dell'adolescente. Manifestò questo disagio in alcuni studi successivi. Successivamente, scusate l'ossimoro, manifestò quasi il contrario: la bellezza

(non sempre ho avuto questa possibilità) sarebbe cambiare troppo il carattere della persona che forse deve vivere con i propri pregi e i propri difetti. Il professor Alberoni

la cosa che fa muovere tutti, secondo Dante anche le stelle, e su qualcosa di ancora più misterioso e complesso soprattutto nel mondo femminile, l'amicizia, la misteriosa miscela di sentimenti che descrive certamente la realtà emotiva più altruistica, più misteriosa,

che in queste poche parole, quelle parole che possono ferire come pietre o essere liberatorie come una poesia di Leopardi o un pezzo

come ha già detto lei, Francesco Alberoni ha avuto un ruolo molto importante per la neonata università di Trento, in particolare per la facoltà di sociologia, ed è in quest'ottica che affronterò questo breve momento commemorativo. Marco Boato, parlamentare di lungo corso, cinque legislature alla Camera e una al Senato, che si laureò proprio con Francesco Alberoni e fu uno dei suoi più stretti collaboratori nella fase di ricostruzione della didattica dell'università di Trento. La fama di Alberoni aveva cominciato ad affermarsi a Trento negli anni caldi dei movimenti di protesta, che avevano avuto il loro epicentro nell'allora Istituto superiore di scienze sociali, dove, per iniziativa del presidente della Provincia autonoma Bruno Kessler, nel 1962, era stato fondato il primo - e all'epoca unico - corso di laurea in sociologia di tutta l'Accademia italiana. Nella primavera del 1968 era stato nominato dal Ministro della pubblica istruzione il Comitato ordinatore di sociologia, con il compito di governare l'Istituto di Trento fino alla costituzione del nuovo consiglio di facoltà. Questo comitato ordinatore era composto dal filosofo Norberto Bobbio, dall'economista Beniamino Andreatta e dallo statistico Marcello Boldrini, che nel 1962, dopo la morte di Enrico Mattei, gli era succeduto alla presidenza dell'ENI. È in questo contesto che il comitato ordinatore, d'accordo con Bruno Kessler che presiedeva il consiglio d'amministrazione dell'istituto, decise di chiamare a dirigere l'Istituto superiore di scienze sociali Francesco Alberoni, che mantenne quell'incarico fino al 1970. Alberoni fino ad allora si era dedicato a studi di sociologia dei consumi e di sociologia dell'immigrazione. A Trento era stato chiamato col compito di governare il rapporto con il movimento studentesco non in chiave repressiva, ma sulla base di una sfida riformatrice. Alberoni prese sul serio questo impegno, dialogando con gli studenti e costruendo insieme a loro l'esperienza totalmente inedita dell'università critica. Verso la fine degli anni Settanta, Alberoni si dedicò ad applicare lo stesso paradigma interpretativo che aveva applicato allo studio dei movimenti collettivi anche ai rapporti interpersonali di coppia, pubblicando nel 1979 il suo libro «Innamoramento e amore», che ebbe un grande successo editoriale, venendo tradotto in venticinque A questo seguirono altri libri e nel 1989 pubblicò anche «Genesi», opera nella quale analizzò i movimenti originati dal cristianesimo, dall'islam e dal marxismo. Dopo sociologia, come ha già ricordato il Presidente di quest'Aula, Alberoni ha insegnato a Catania, a Milano, allo IULM e ha avuto numerosi incarichi in consigli di amministrazione. Di lui resta una bibliografia imponente e molto varia, anche se i *mass media*, alla notizia della sua scomparsa, hanno ridotto la sua biografia intellettuale soltanto allo stereotipo del sociologo dell'amore, ma nel quadro della storia del pensiero sociologico, non solo italiano, il suo apporto più significativo e duraturo resta proprio la sua analisi e interpretazione sistematica dei movimenti collettivi, che cominciò ad elaborare negli anni, ormai assai lontani, del suo impegno alla facoltà di sociologia di Trento. Non è semplice spiegare alle nuove generazioni il clima di quegli anni, la voglia di stabilire canali di dialogo e confronto tra la Trento di allora, i giovani politicizzati, e un'istituzione universitaria che in alcune sue componenti opponeva una strenua resistenza alle spinte riformatrici. Concludo dicendo che fu un lavoro faticoso, ma anche entusiasmante, perché aveva come punto di contatto la cultura, a conferma che il sapere è il nostro antidoto contro i pregiudizi e per avvicinare i diversi, quel sapere che Francesco Alberoni ha coltivato per tutta la sua vita: il suo lascito più grande, la sua eredità.

ai parenti, ai familiari tutti, ai figli del sociologo Francesco Alberoni anche da parte del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe.

quella che stiamo ricordando è una figura importante, un sociologo, un accademico, un giornalista, uno scrittore, un uomo impegnato anche nelle istituzioni,

Mi piace, però, sottolineare quello che lei Presidente ha detto anche all'inizio del suo discorso, ovvero l'empatia di Francesco Alberoni. Per chi, come quelli della mia generazione, ha letto

Un uomo, come è stato definito, prima di tutto con grandi doti umane, un uomo empatico che ha saputo parlare un linguaggio, come lei ha ben sottolineato, semplice, quindi universale,

Come è stato ben sottolineato, lo ricordiamo certamente per alcuni aspetti, in modo particolare è stato il primo studioso a scrivere di sociologia dei consumi e anche il più importante studioso internazionale dei movimenti collettivi, ma soprattutto ha studiato per tutta la sua vita professionale l'innamoramento, le dinamiche dell'amore, il tema dell'amicizia, del divismo.

«Innamoramento e amore» del 1979, tradotto in ben 24 lingue, tanto da valergli il riconoscimento a livello mondiale come sociologo della fenomenologia dell'amore, l'indagatore dei misteriosi meccanismi per cui nasce il legame tra due persone che si scelgono. Ci sono tanti altri suoi libri di cui potremmo parlare, che hanno segnato sicuramente una fase importante dal punto di vista sociologico del periodo storico che abbiamo vissuto. Concludo, signor Presidente, ricordando una frase tratta proprio dal libro «Innamoramento e amore», che credo sia anche consona a quest'Aula.

è una forza immensa, capace di fondare Nazioni, di deviare le vite delle persone, di cambiare la storia». «L'amore tende a separare la legge dalla persona; vuol instaurare altre leggi, altre norme». Mi sembra un modo anche bello per poterlo ricordare in quest'Aula così importante. *(Applausi)*.

poche parole per ricordare oggi la figura di un grande uomo di cultura e di un grande divulgatore, capace come pochi di narrare le dinamiche dell'innamoramento e dell'amore, come è già stato detto da alcuni colleghi, ma in modo da riuscire a raggiungere chiunque, utilizzando parole comprensibili ed immediate. Probabilmente un lessico semplice e di uso quotidiano, ereditato dalla sua infanzia nella provincia di Piacenza e filtrato da anni di studi universitari in medicina prima e poi di ricerche psicologiche, sociologiche e filosofiche. Essere stato allievo di padre Agostino Gemelli, che aveva fondato l'università Cattolica del Sacro Cuore, gli diede certamente quell'impulso a diventare, come lui stesso si definiva, un imprenditore culturale. Infatti partecipò alla creazione e costruzione dell'Università di Scienze e Comunicazione (lo IULM di Milano), di cui fu per anni professore e poi rettore. Anni dopo, come presidente del Centro sperimentale di cinematografia di Roma, diede anche qui nuova vita alla principale scuola di cinema italiana. È stato senza dubbio una figura di intellettuale non schierabile: antifascista durante il fascismo e poi simpatizzante della destra della *premier* Meloni senza infingimenti, senza nascondere nulla, con la semplicità che un intellettuale impegnato nella vita e impegnato nella creazione di ogni cosa che lo circondasse e che incontrasse non poteva non avere. Non poteva venir meno al dovere di un impegno ad ogni attimo della propria vita e a ogni angolo che si incontrasse di impegno sociale e civile, in questo caso anche politico. La dimostrazione di quanto fosse amato e seguito sta nei milioni di copie vendute dei suoi libri. Non dobbiamo certo né inventarlo, né citarlo più di tanto; lo sappiamo tutti. Sono testi che tra l'altro sono stati tradotti in venticinque lingue, a dimostrazione della facilità di comprendere argomentazioni che lui è stato capace di rendere alla portata di tutti. La sua storia personale ed intellettuale ce lo fa ricordare come un testimone attento della vita culturale e civile italiana. Ci ha lasciato dopo una vita carica di traguardi e di successi, ma il suo insegnamento - ci sentiamo di dire - è oggi quanto mai attuale.

la nostra Assemblea oggi, con la prima seduta del 2024, si apre con la commemorazione di due uomini illustri, che hanno lasciato veramente un segno indelebile nella nostra storia e nella nostra cultura. Il professor Francesco Alberoni, che è venuto a mancare lo scorso agosto, è stato un grande sociologo, un intellettuale, un innovatore che ha dedicato la sua vita alla ricerca della conoscenza, all'analisi e alla comprensione dei fenomeni sociali complessi, dimostrando così una rara capacità nel renderli accessibili Ha raccontato e interpretato l'Italia dei primi anni Sessanta praticamente fino ai giorni nostri. Il professor Alberoni ha osservato la società e i suoi cambiamenti, studiandone principalmente due aspetti fondamentali: da una parte la nuova industrializzazione, con il peso della fabbrica e la presa di coscienza politica dei lavoratori e poi anche dei giovani universitari; dall'altra parte ha osservato lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, *in primis* la televisione, e l'avanzare dei consumi di massa. Ha seguito l'evolversi di questi elementi in trasformazione con un occhio particolare rivolto alle giovani generazioni, che erano al centro di cambiamenti ancora più imponenti. Proprio a partire dall'analisi dei movimenti studenteschi, delle proteste e della rivolta del '68 è nato il saggio «Movimento e istituzione», del 1977, in cui l'analisi dei movimenti collettivi, che fino a quel momento era mancata, è arrivata ad individuare la condizione nascente, secondo il professor Alberoni, lo stato nascente all'interno dei movimenti di massa. Ha così centralizzato quello che era un momento di svolta, dove l'innamoramento per le idee, la focalizzazione del gruppo su uno o più *leader*, la comunicazione delle idee e la loro diffusione arrivavano a fondersi e a far nascere così il movimento. In una delle sue ultime interviste ha ricordato, con la capacità comunicativa che lo contraddistingueva, come è nata poi la sua fama di studioso dei movimenti e questa sua figura di sociologo che capisce i movimenti.

Le attività del professor Alberoni hanno rappresentato veramente un ponte fra l'ambito accademico e la sfera sociale esterna, ispirando così a comprendere e affrontare dinamiche sociali in modo anche più consapevole. Il suo contributo nella divulgazione ha favorito una connessione tra le teorie sociologiche e la stessa azione politica, arricchendo il dibattito pubblico con una comprensione più approfondita delle sfide sociali. Alberoni è stato anche un visionario. Un suo libro del 2021, «Il rinnovamento del mondo», racconta la storia che si svolge tra due date: la prima è quella della caduta del Muro di Berlino e la seconda è quella in cui inizia l'epidemia da Covid-19. Con la prima termina la divisione del mondo in due blocchi ideologici, il mondo atlantico e quello sovietico, e incomincia un processo di globalizzazione in cui scompaiono le frontiere tra gli Stati, scompare l'immagine di un nemico e tutto appare uniforme. La seconda data cade quando questo processo ha fine. Nei suoi interventi successivi aveva anche evidenziato come, dopo trent'anni di globalizzazione, con la scomparsa dell'identità ci sarebbe stato un ritorno delle identità nazionali e della Nazione e sarebbe emerso un conflitto per il potere mondiale, prefigurando l'ingresso di una nuova epoca, quella degli Stati combattenti, nella quale diverse potenze auspicano il potere mondiale. L'eredità del professore Alberoni vive attraverso le sue opere, che continueranno ad ispirare e guidare non solo le future generazioni di ricercatori e gli appassionati di sociologia, ma tutti noi. Il suo spirito vivace, le sue idee e le sue opere sono veramente un tesoro di saggezza e ispirazione per comprendere davvero le dinamiche sociali complesse.

Presidente, ringrazio il mio Gruppo per il privilegio che mi ha assegnato di poter ricordare in quest'Aula, come hanno fatto già altri colleghi e come ha fatto lei stesso, la figura di Francesco Alberoni. Il suo spessore, il suo eclettismo e la sua multidisciplinarietà culturale sono già stati ben delineati sia nella sua introduzione che da tanti altri interventi. Per questo voglio solo tratteggiare alcuni elementi della sua figura, che ne hanno giustamente fatto una delle personalità di maggiore rilievo della seconda parte del Novecento fino al ventennio che abbiamo attraversato di questo nuovo secolo. Abbiamo tutti noi ammirato sempre in Francesco Alberoni la sua volontà, la sua capacità, la sua condizione naturale di essere empatico con coloro ai quali lui rivolgeva i suoi scritti, i suoi studi, i suoi lavori. La divulgazione per lui non era un'opinione; non lo era nella divulgazione della ricerca e dei suoi studi, e tutta la sua bibliografia è stata tesa a parlare non soltanto ai colleghi, agli addetti ai lavori, al mondo accademico, ma anche alla società. In questo senso non è stato un sociologo *in vitro*, ma è stato davvero un ricercatore e un analista delle mutazioni dei comportamenti sociali sulla base di verifiche fatte sul campo. I suoi numerosi incarichi che sono stati ricordati confermano anche questo. Molti sono stati gli spunti originali che ne hanno fatto una figura di spessore non solo italiano. Ad esempio - mi pare forse lo ricordasse poco fa la senatrice Stefani della Lega - in «Statu nascenti» fornì un'interpretazione dei movimenti del 1968 basata sull'idea di condizione nascente, cioè intesa come un momento nel quale le idee e la comunicazione si fondono dando origine a un movimento collettivo. Scopre cioè che le proprietà dello stato nascente esistono, per analogia, anche in un fenomeno apparentemente diversissimo come l'innamoramento. Ha ragione il senatore Patton: non si possono ridurre la complessità e lo spessore di Francesco Alberoni a innamoramento e amore, ma è anche vero che l'opera sua più nota e più diffusa a livello anche internazionale ha marcato la cultura e il costume italiano. Pensate che, nel 1979, quando uscì, quest'opera fu presentata 1979, quando uscì, quest'opera fu presentata anche al Festival nazionale dell'Unità: un successo immediato. Lui rivoluzionò anche lo stile sociologico, arrivando a usare il linguaggio tipico della letteratura amorosa dei giornali più popolari. popolari. Era il tempo in cui dominavano le ideologie e due straordinari personaggi, Gianni Vattimo ed Enrico Filippini, su «Repubblica» mossero critiche anche - critiche culturali, naturalmente - al lavoro di Alberoni. Per esempio, Vattimo, su «La Stampa», parlò di un mito di fatto irrealizzabile. Secondo Vattimo il mito irrealizzabile riguardava l'idea che l'amore allo stato nascente non possa avere la forza dirompente dei movimenti rivoluzionari, cosa che invece Alberoni assegnava appunto all'innamoramento. Filippini, su «Repubblica», ugualmente fece analisi molto critiche, paragonando in qualche modo in maniera provocatoria - lo scritto di Alberoni a Mike Bongiorno e alle consulenti del cuore note ai giornali "femminili" dell'epoca. In conclusione, c'è un elemento che vorrei rilevare, perché ha una grande attualità. analizzò molto il fenomeno del divismo nella società contemporanea: un fenomeno che negli anni Settanta definiva l'*élite* senza potere, cioè in pratica personalità della cultura e dello spettacolo che non avevano potere istituzionale o potere economico, ma che tuttavia influenzavano influenzavano molto l'opinione pubblica. In sostanza, accanto al potere dell'*élite* c'era anche il potere di personalità i cui gesti influenzavano la società e le persone. Il divo veniva definito colui che era dotato di proprietà carismatiche. Ecco, per Alberoni - e questo è davvero profetico Presidente - dalla fusione del mondo del divo con quello del potere tradizionale poteva e può nascere un grave pericolo per le società democratiche: il pericolo che il carisma del politico si trasferisca al divo, i cui comportamenti sono spesso discutibili Grazie

curioso, appassionato, originale e coraggioso: sono le caratteristiche di un uomo e di uno studioso che ha cambiato la storia delle scienze sociali nel nostro Paese. Con la scomparsa di Francesco Alberoni abbiamo perso una figura di enorme *standing*, un uomo che con le sue riflessioni ha dato lustro all'Italia e contribuito alla formazione umana di tutti noi. Con la sua opera di sociologo, accademico e scrittore, ha indagato i movimenti collettivi della nostra società. Con occhio attento ha analizzato profondamente la partecipazione politica, il nostro modo di comunicare e di relazionarci tra di noi. Ha generato una forza innovatrice e un pensiero critico capaci di contribuire al progresso e all'ammodernamento culturale dell'Italia del Dopoguerra. Ha contribuito a traghettare il nostro Paese nell'età moderna con eleganza e fruibilità, coniugando la raffinatezza dell'intellettuale alla comprensibilità dell'uomo mai distante ma immerso nella società che descriveva. Mi piace ricordarlo attraverso due concetti a lui cari, il primo dei quali è quello della *leadership*. Diceva il professore che il *leader* è prima di tutto il custode della meta, colui che ricorda e indica a tutti dove si deve andare e controlla che la rotta venga mantenuta. Deve trasmettere a ogni livello dell'organizzazione il senso della missione, il significato del compito e il senso del dovere. Solo chi è mosso da una visione può fare ciò che gli altri non riescono nemmeno a pensare o immaginare. Il secondo concetto riguarda l'amore e la bellezza. Diceva il professore: «E, quando cogliamo la bellezza di un paesaggio o di un'opera d'arte con lei, abbiamo una esperienza che è in qualche modo affine al rapimento amoroso. In quell'istante è come se cadessero le barriere che ci isolano dal mondo e l'essenza dell'oggetto irrompe, si impossessa di noi. Come nell'amore quando entriamo in contatto diretto con la natura profonda dell'altro, ne cogliamo l'incredibile stupefacente e unicità.». Con prova di coraggio e lungimiranza, nel 2019 il professor Alberoni decise di candidarsi con Fratelli d'Italia; una candidatura realmente al servizio del Paese, lontana da dogmi ideologici, frutto della stima verso una donna, una giovane *leader*, ambiziosa e controcorrente, come Giorgia Meloni, lontano dallo *status quo* del mondo politico di quel periodo. Non fu eletto, ma quella scelta coraggiosa, per certi versi rivoluzionaria per un accademico che non aveva certo bisogno della politica per esistere, contribuì a costituire una forza propulsiva, in grado, qualche anno dopo, di scompaginare il sistema politico italiano e portare Fratelli d'Italia a esprimere la prima donna Presidente del Consiglio del nostro Paese. Il nostro Gruppo parlamentare e il Paese intero non possono che esprimere gratitudine al professor Alberoni, per aver dimostrato come, con l'impegno, il senso critico e il proprio coraggioso esempio, sia possibile contribuire a costruire il futuro di una società migliore, più aperta, democratica e accogliente. così conclusi gli interventi commemorativi del professor Francesco Alberoni. Mi resta solo, nel ricordare ancora una volta l'amico Francesco, di ringraziare i familiari per la loro presenza qui tra noi in Senato. Grazie ancora di cuore.

Colleghe senatrici, colleghi senatori, ricorre proprio oggi il ventesimo anniversario della scomparsa del senatore a vita Norberto Bobbio, una delle menti più influenti della nostra epoca e del pensiero democratico. Filosofo, giurista, storico, politologo e accademico italiano, attraverso le sue opere Norberto Bobbio ha accompagnato lo sviluppo della nostra comunità nazionale, nel solco di ideali di partecipazione, pluralismo e dialogo. La sua lunga carriera accademica si è spesso intrecciata con un'instancabile impegno civico e politico; un impegno culminato, nel 1984, con la nomina a senatore a vita da parte del presidente Sandro Pertini per altissimi meriti in campo sociale e scientifico; un ruolo che il senatore Norberto Bobbio ha ricoperto per ben sei legislature, con rigore e passione, diventando un irrinunciabile punto di riferimento per tante generazioni di politici, di parlamentari, donne e uomini dello Stato. Le sue analisi e le teorie da lui elaborate, i suoi insegnamenti come ha ricordato oggi anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella - sono e saranno oggetto di approfonditi studi nei più prestigiosi luoghi di cultura. Ricordarne la figura oggi significa soffermarsi a riflettere sui suoi insegnamenti e in particolare su come egli considerasse la democrazia cardine irrinunciabile di libertà, pace, giustizia e tutela dei diritti; una democrazia che egli ci invita a difendere come ideale morale e politico. In memoria del senatore a vita Norberto Bobbio, invito, pertanto, l'Aula a osservare un minuto

essere chiamati a parlare per cinque minuti per ricordare Norberto Bobbio è uno di quegli incarichi impossibili che qualche volta la politica e la vita ti offrono.

al contrario di quello che accade di solito, non sia meno sentita. Il passaggio del tempo non sta attenuando il ricordo della sua opera e del suo pensiero, ma

In un'epoca nella quale il messaggio politico si è completamente ipersemplificato, in un momento nel quale il pensiero si è ridotto spesso a un telegramma, allo spazio di un *tweet*, a 140 caratteri, il ragionamento di Bobbio ci invita invece alla complessità, alla profondità, al

debba essere sempre svolto all'interno di un grande rispetto reciproco. È questa una delle ragioni per le quali io credo che oggi ci manchi. la nettezza - da un lato - delle posizioni di Bobbio che, certo, non faceva sconti; che difendeva la forma repubblicana e l'antifascismo con una chiarezza che definirei inossidabile che non consentiva sconti; e - dall'altro lato

e, quindi, di essere capaci di discutere le differenze in quel confronto reciproco che era comunque di beneficio all'intera comunità perché l'avrebbe fatta crescere nel suo insieme. Penso che questo oggi sia ciò che che più ci manca di Norberto Bobbio. Oggi, in un momento nel quale perdiamo il senso di alcuni valori repubblicani

a chi nella sua attività politica ha provato a perseguire l'approfondimento più che lo *slogan*. Mi vengono in mente, ad esempio, alcuni dilemmi che nell'opera di Bobbio vanno a confrontarsi. Pensiamo ad esempio al confronto tra l'uguaglianza e la libertà: due polarità intorno alle quali le più nobili famiglie politiche si sono esercitate. Sono necessariamente uguaglianza e libertà valori contrastanti per i quali ci si può schierare alternativamente? Stiamo con la libertà o stiamo con l'uguaglianza? Oppure il confronto e l'apertura, la tolleranza - una parola che a me non piace molto, perché penso che si tollerano gli insetti e non le persone - l'inclusione e il rapporto di rispetto reciproco conoscono dei confini o sono illimitati? Si può essere tolleranti con gli intolleranti? Si può accettare, nel nome dell'apertura, che si vada anche al di là di quei cardini fondamentali che devono essere la la base del nostro contratto sociale? Ecco io credo che il pensiero di Norberto Bobbio, questo tipo di esercizio, manchi grandemente alla politica contemporanea. Penso che ci farebbe molto bene recuperarlo e credo che, a distanza di vent'anni, la sua assenza e il suo vuoto si sentano paradossalmente - come dicevo all'inizio - forse più ancora di quanto si sentirono nel momento in cui ci lasciò. Signor Presidente, per la mia generazione, quando eravamo giovani militanti di sinistra, Norberto Bobbio è stato l'emblema stesso di quella grande cultura liberale italiana che, pur nelle differenze, intratteneva con la corrente di pensiero socialista e marxista un rapporto di interlocuzione e dialogo. Era Bobbio il gigante del pensiero liberale che negli anni Ottanta, evidenziando la sua disillusione per alcune involuzioni della democrazia italiana, confessava di aver nutrito grandi e deluse speranze solo in tre occasioni, una per decennio: dopo la sconfitta della legge truffa nel 1953, al momento della nascita del primo centrosinistra nel 1964 e poi con il grande balzo elettorale del Partito Comunista Italiano nel 1975. Bobbio era un liberal democratico, come oggi si proclamano quasi tutti, e un'azionista, ma specificava che, pur non essendo mai stato comunista, aveva sempre considerato i comunisti - o almeno i comunisti italiani - non come nemici da combattere, ma come interlocutori di un dialogo sulle ragioni della sinistra. Dunque, era anche per noi un punto di riferimento e spesso un maestro. Con la cultura assembleare e con le istanze di democrazia diretta che, a partire dal 1968, segnarono in Italia il dibattito politico, dunque la nostra cultura, Bobbio era certamente critico, ma non perché non ne condividesse le spinte e le ragioni di fondo: riconosceva anzi che la frontiera della democrazia fosse la sua estensione dalla sfera della politica a quella del sociale. Segnalava la necessità di estenderla a quei luoghi in cui il potere si esercitava ancora solo dall'alto in basso, in particolare nei luoghi di lavoro e nella pubblica amministrazione. Indicava però una strada diversa per raggiungere quel traguardo: non uno stravolgimento delle regole del gioco, ma la loro estensione agli ambiti dai quali erano ancora banditi. Per tutta la vita Norberto Bobbio ha insistito nel sottolineare che la democrazia è soprattutto una questione procedurale che attiene essenzialmente alle regole del gioco. Con le sue stesse parole, è «un metodo per prendere decisioni collettive»: tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente e la decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. In questa formula non c'è nulla di minimalista o di scolastico. A muovere Bobbio era invece la convinzione appassionata che la democrazia non è una conquista data una volta per tutte e che nulla sia più pericoloso nel ritenerla tale. Diceva inoltre che i nostri padri erano democratici ottimisti e che noi siamo e dobbiamo essere sempre democratici in allarme. La La sua insistenza sulla centralità delle procedure e la sua continua analisi del funzionamento delle regole democratiche, puntigliosa e lucidissima, erano nel suo modo di essere sempre in allarme e di tenere tutti noi democratici, liberali o socialisti che fossimo, sempre sul chi vive. Quel dibattito sembra oggi preistoria, lontanissimo. Dalla morte del senatore a vita Norberto Bobbio in poi, vent'anni fa, abbiamo assistito a un progressivo svuotamento di senso di quella democrazia, sulle cui sorti ci esortava a restare sempre vigili. La partecipazione è stata ridotta progressivamente a un simulacro e la rappresentanza - principio sul quale aveva scritto alcune delle sue pagine più incisive - spogliata di quasi ogni significato. Sono in campo - come sappiamo - proposte di riforma costituzionale che, almeno a mio parere, implicherebbero il fortissimo rischio di degenerazione democratica, in una sorta di autocrazia autocrazia elettiva. Per questo oggi più che mai è necessario ricorrere al pensiero di Norberto Bobbio e adoperarlo per quello che voleva essere: una mappa strategica per difendere, ma anche per allargare, la nostra democrazia. Signor Presidente, colleghi senatori, dopo il professor Alberoni, tocca a me oggi commemorare un altro socialista. Norberto Bobbio è stato un pensatore influente che ha modernizzato la cultura politica nazionale, un filosofo del diritto che ha saputo arricchire con la sua produzione scientifica l'evo contemporaneo; un intellettuale che nel lungo tragitto del Novecento, segnato dalle dinamiche distruttive dei totalitarismi e delle guerre mondiali, non ha mai smarrito la bussola dei diritti e della libertà, nutrimento di impegno civile e morale.

Bobbio amava definirsi uomo del dubbio e del dialogo, continuamente portato a farsi domande, a sospendere i giudizi, a mettere in discussione gli approdi, a investigare le ragioni altrui per coglierne fino in fondo l'essenza. Osservatore attento e al contempo preoccupato, egli rifletteva sul futuro, oltre che sul concetto stesso di democrazia, da tenere saldamente legato alla giustizia sociale; sulle sfide molteplici che ne fiaccavano lo spirito e sul ruolo degli uomini di cultura, per rafforzarne gli argini. Egli soleva ripetere: «Cultura significa misura, ponderatezza, circospezione: valutare tutti gli argomenti prima di pronunciarsi, controllare tutte le testimonianze prima di decidere, e non pronunciarsi e non decidere mai a guisa di oracolo da quale dipenda, in modo irrevocabile, una scelta perentoria e definitiva». quest'Aula si celebra oggi il ventesimo anniversario della scomparsa di un uomo di statura capace di rompere gli schemi e sfidare il conformismo, pagandone le conseguenze pur di non rinunciare al bisogno di comprensione e al gusto o al dovere della verità. Fra le innumerevoli pagine della biografia di intellettuale impegnato, ne cito una, quella che Bobbio compose negli anni Settanta del secolo scorso, quando la visione marxista della società andava imponendosi come un valore acquisito. Le sue argomentazioni, pubblicate sulle colonne della rivista «Mondoperaio», una delle riviste intellettualmente più vivaci della galassia socialista, seminarono dubbi sull'esistenza di una dottrina marxista dello Stato, squarciarono il velo delle ipocrisie segnando l'avvio di un processo di rinsavimento culturale e politico dell'area social-riformista. Interprete e critico autorevole della Repubblica dei partiti, Bobbio accompagnò con una sorta di amaro disincanto il passaggio a una diversa fase della storia politica nazionale, nel tornante conclusivo del XX secolo. Egli certamente si schierò contro le degenerazioni sistemiche, ma prese pure di petto le tendenze alla disgregazione particolaristica della società civile in nome della quale si esaltavano le virtù salvifiche dell'antipolitica. Vi è traccia di questo approccio nell'editoriale pubblicato sulla prima pagina del quotidiano «La Stampa» il 20 gennaio del 1993. «La prima Repubblica» - scrive Bobbio - «è proprio finita. Non lo dico, come la maggior parte degli italiani, con un sospiro di sollievo o addirittura con aria di trionfo. Lo dico con un senso di amarezza perché una conclusione così miseranda è l'espressione del fallimento di tutta intera la nazione, e non solo della classe politica che è ormai continuamente e rabbiosamente messa sotto da parte di coloro che per anni l'hanno sostenuta e le hanno offerto il consenso necessario per governare. Come paese democratico, come Stato di liberi cittadini, abbiamo fatto, bisogna riconoscerlo, una pessima prova». Norberto Bobbio, come gli altri intellettuali del secolo scorso, ha legato il suo nome a un processo storico di contaminazione feconda tra politica e cultura, rivendicando certo l'autonomia del sapere dai condizionamenti del potere, ma riconoscendo l'importanza di un legame da cui poteva trarre giovamento non solo il profilo identitario della Nazione, ma pure gli sforzi tesi a definire le categorie interpretative per leggere la modernità. la ricchezza del nostro Paese non è nel benessere economico. La vera ricchezza è nell'eredità culturale che abbiamo ricevuto dai nostri intellettuali, dai nostri filosofi, dai nostri poeti. È la cultura che nutre la nostra anima. E devo dire che Bobbio ci ha lasciato una grande eredità, un patrimonio culturale fatto di valori che riflettono la sua natura di uomo del diritto, di umanista. È inevitabile, nel ricordare Bobbio, farci tornare alla mente il suo amore per i diritti umani, il suo amore per la democrazia e soprattutto il suo amore per il dialogo democratico.

il suo pensiero e la sua vita sono stati caratterizzati dall'incessante ricerca volta a trovare una mediazione tra le varie opinioni in campo. Questo forse è stato il suo più grande insegnamento. Uno dei suoi pensieri che più mi ha colpito è mettersi sempre, nei confronti dell'altro, in un atteggiamento che deve farci un po' rinunciare all'idea di essere depositari di una verità assoluta. Scriveva che tra la verità e la non verità c'è sempre spazio per una verità da sottoporre a continuo revisionismo. E ci avvertiva anche di un fatto: dobbiamo credere nelle buone ragioni, perché, se smettiamo di farlo, lì inizia la violenza. Scusate, colleghi, c'è un po' di brusio che mi distrae. Pensate quanti conflitti e quante guerre sono nati perché a monte è mancato questo spirito di dialogo. Un'altra cosa importante: quando Bobbio ci parla della necessità di dialogare e di rispettarsi, in realtà ci fa capire che questo non serve soltanto come un atteggiamento di rispetto dell'altro, perché aprirsi al dialogo significa anche arricchire noi stessi. Tutte le volte che noi nell'avversario immaginiamo di vedere un nemico ci stiamo sottraendo a una delle nostre opportunità, l'opportunità di aprirsi a delle nuove consapevolezze. consapevolezze. Vorrei citare le parole di un altro intellettuale del nostro tempo, che in qualche maniera fanno eco alle parole di Norberto Bobbio. Questo intellettuale diceva: «Dovremmo ospitare il sospetto che l'altro sia abitato dalla verità». Proviamo a soffermarci su questa espressione "abitato dalla verità". È un po' come richiamare l'idea che il nostro pensiero stia maturando nel nostro mondo interno: il contatto con l'altro ci costringe a confrontare due mondi interni, il nostro mondo interno da cui si genera il pensiero. A volte proiettiamo sull'altro qualcosa che non siamo in grado di accettare in noi stessi. Abbiamo quasi paura di guardare quella parte del nostro mondo interno che ci fa in qualche maniera mettere nel dubbio un'idea. La difficoltà di dialogare non dipende dal fatto che abbiamo idee diverse o che abbiamo colori politici diversi. Il più grande ostacolo al dialogo democratico e al confronto, anche in quest'Aula, è dato dalle nostre paure e dai nostri pregiudizi. Norberto Bobbio ci mette in guardia da questo e ci dice che, per entrare in contatto con l'altro, dobbiamo spogliarci di questi pregiudizi, dobbiamo essere nudi per poter affrontare il dialogo. Questo però - attenzione - non vorrei che venisse interpretato come l'idea di un relativismo culturale. Tutt'altro: è semplicemente acquisire la consapevolezza della complessità. Noi viviamo in una realtà in cui ciascuno di noi deve deve credere nei suoi principi e far valere i suoi principi. L'importante è che questi principi non si trasformino nella presunzione di una verità assoluta, che non diventino dei dogmi.

e chi crede di essere depositario della verità assoluta. prendere questa parte della sua eredità e imparare soprattutto a rispettarci gli uni con gli altri. Se impariamo a rispettarci tra di noi, è lì che stiamo davvero rispettando quella popolazione che ciascuno di noi in quest'Aula sta rappresentando. *(Applausi)*.

difficile sintetizzare in un breve intervento il ricordo di una figura così importante per la storia e la cultura italiana. Come ha scritto Michelangelo Bovero: «Non ogni studioso è anche un intellettuale. Lo studioso cerca di comprendere, di interpretare, di spiegare il mondo; l'intellettuale giudica, valuta, cerca di influenzare atteggiamenti e comportamenti». Ecco, Bobbio era uno studioso e un intellettuale. Come disse lo stesso Bobbio commentando Feuerbach: prima di cambiare il mondo, bisogna interpretarlo. Quindi bisogna anche essere studiosi e bisogna conoscerlo. Dicevo che è impossibile sintetizzare in un intervento un pensiero così complesso. Sarebbe ovvio e scontato, per un leghista come me, ricordare il Norberto Bobbio sostenitore della causa federalista. Ci concentriamo invece su un altro aspetto: sulla lettura o, per meglio dire, la rilettura che Bobbio ha fatto della Resistenza. Come il filosofo Derrida, Bobbio scava la parola Resistenza fino a toccare le vertigini di un passato che non passa, fino ad arrivare al significato più profondo, e definisce la Resistenza una guerra civile. Quando lo fece, suscitò parecchio scalpore. Lo fece ad esempio nel libro «Dal fascismo alla democrazia». Già il titolo di questo saggio molto importante dice tutto. La Resistenza è una cesura netta tra la non democrazia e la democrazia. Ma Norberto Bobbio, liberale socialista, non è mai stato divisivo. La definizione stessa di Resistenza come guerra civile, di guerra di italiani contro italiani, è non un giudizio di valore, ma una constatazione, un dato di fatto. Non è divisiva la definizione delle tre guerre civili così le descrive nel testo, anche questo molto interessante, «Sulla guerra civile», scritto con Claudio Pavone - ossia la guerra patriottica contro l'esercito nazista invasore, la guerra civile contro la dittatura fascista, la guerra di classe per le emancipazioni sociali: tre guerre che non necessariamente sussistono contemporaneamente nei singoli partecipanti alla Resistenza. Alla fine, quello che resta del pensiero di Bobbio sul concetto di Resistenza, dopo la Resistenza, dopo la guerra civile, è questa cesura: dal fascismo alla democrazia, dalla non democrazia alla democrazia e in mezzo c'è la guerra civile. E così la descrive, la descrive, la racconta profondamente e semplicemente Cesare Pavese: «Ora che ho visto cos'è guerra, cos'è guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero». Signor Presidente, colleghi e colleghi, siamo oggi chiamati a onorare, nel ventennale della sua morte, un grande italiano. Come ha avuto modo di ricordare il Presidente della Repubblica: «La Repubblica, grata a Norberto Bobbio per aver illustrato la Patria con i suoi altissimi meriti nel campo scientifico, lo volle senatore a vita». Studioso dei fenomeni che hanno dato impulso alle più significative vicende storiche del secolo scorso, Norberto Bobbio, ha elaborato dottrine che costituiscono una preziosa eredità per la coscienza civile europea e italiana. Nasce nel 1909 a Torino, dove frequenta il liceo D'Azeglio e incontra Ginsburg, Foa, Pavese. Sempre a Torino si laurea in giurisprudenza e poi in filosofia. A Torino muore nel 2004, dopo aver insegnato a Camerino, Siena, Padova e poi Torino, prima filosofia del diritto e poi, dal 1972, filosofia della politica. Diritto e filosofia: nel passaggio all'insegnamento dall'uno all'altra si vogliono vedere due fasi della sua vita intellettuale, ma si esprime anche quell'intimo nesso che ha sempre legato, nel pensiero di Bobbio, diritto e democrazia, teoria del diritto e filosofia politica. Norberto Bobbio fu un filosofo militante, come egli stesso ebbe a dire di Cattaneo nel saggio a lui dedicato. Nominato senatore a vita nel 1984, aderì come indipendente al Gruppo socialista; poi, dal 1991 al Gruppo Misto e infine dal 1996 al Gruppo parlamentare del Partito Democratico della Sinistra, poi Democratici di Sinistra. Del resto, già durante la Seconda guerra mondiale, Norberto Bobbio era entrato a far parte del Partito d'Azione e dal 1942 aveva partecipato alla Resistenza, prima a Padova, poi a Torino. lontano da un'idea di apoliticità dell'Accademia, ma allo stesso tempo lontanissimo dalla politicizzazione che riduce la filosofia a un servizio pubblico. Del resto, sul ruolo degli intellettuali e il loro impegno ebbe importanti discussioni, anche polemiche, con Togliatti e Della Volpe, esprimendo una concezione del ruolo della cultura che si ritrova in «Politica e Cultura», appunto, del 1955. Bobbio, nel Dopoguerra, ha sprovincializzato la cultura italiana. L'ha aperta a nuovi orientamenti filosofici, dalla logica alla filosofia della scienza, alla sociologia, alla scienza politica. Luigi Ferrajoli lo ha definito «filosofo della ricostruzione» dopo la catastrofe della guerra e della chiusura intellettuale della dittatura. In Bobbio ragione, diritto e democrazia si legano. La democrazia è costruzione giuridica e il diritto è lo strumento per garantire la democrazia e la pace. Scrive Scrive egli stesso ne «L'età dei diritti» che il riconoscimento e la protezione dei diritti dell'uomo stanno alla base delle Costituzioni democratiche moderne. La pace è a sua volta il presupposto necessario per il riconoscimento e l'effettiva protezione dei diritti dell'uomo nei singoli Stati e nel sistema internazionale. Bobbio fu l'uomo del socialismo liberale in un confronto serrato con la tradizione marxista e con lo stesso Partito Comunista. Bobbio sottolineava l'importanza delle istituzioni liberali e della democrazia politica, a cui dedicò, nel 1984, il saggio «Il futuro della democrazia». Ma Bobbio è anche il pensatore delle dicotomie - come ci ha ricordato oggi Zagrebelsky - ma non delle chiusure dogmatiche: destra e sinistra, fascismo e antifascismo, intolleranza - tolleranza. l'uomo che si chiede, di fronte alla vittoria delle democrazie nei confronti del comunismo storico, come la democrazia possa affrontare i problemi da cui la sfida del comunismo era nata, le grandi questioni sociali, le diseguaglianze, la democrazia sociale. In un'intervista a Bosetti del luglio del 1989, poco prima della caduta del muro, che si intitola appunto, non a caso, «Adesso la democrazia è sola», il grande tema è quello della giustizia sociale nel mondo e come perseguirla insieme alla libertà. Nel 1994, quando emergono, col crollo del sistema dei partiti, nuovi attori della vita pubblica, Bobbio pubblica «Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica» allora e oggi imprescindibile. E lo fa anche con un'annotazione personale che qui voglio citare e chiudo: «mi sono sempre considerato un uomo di sinistra e quindi ho sempre dato al termine Sinistra una connotazione positiva, anche ora che è sempre più avversata, e al termine Destra una connotazione negativa, pur essendo oggi ampiamente rivalutata. La ragione fondamentale per cui in alcune epoche della mia vita ho avuto qualche interesse per la politica, o con altre parole ho sentito se non il dovere, parola troppo ambiziosa, l'esigenza di occuparmi di politica e qualche volta, se pure più raramente, di svolgere attività politica, di fronte allo spettacolo delle enormi diseguaglianze, tanto sproporzionate quanto ingiustificate, tra ricchi e poveri, tra chi sta in alto e chi sta in basso nella scala sociale, tra chi possiede potere, vale a dire la capacità di determinare il comportamento altrui, sia nella sfera economica sia in quella politica e ideologica, e chi non ne ha». Sono parole importanti oggi che la passione verso l'uguaglianza sembra essersi raffreddata, ma che tornano più che mai tutte le ragioni per un impegno in questo senso e che fanno di Bobbio un punto di riferimento essenziale.

anche se ovviamente ristretta, rievocazione della sua figura, bisognerebbe rifarsi al discorso che l'allora Presidente del Senato, Marcello Pera, fece in tale occasione. Oggi io non posso certo pensare di avvicinarmi a quanto il professore, nonché presidente Pera disse in quell'epoca. Norberto Bobbio è stata una figura di straordinario prestigio nella nostra vita culturale. Egli avrebbe potuto restare in ambito intellettuale, accademico, senza senza sporcarsi le mani nel confronto politico, nel senso di confronto di idee, naturalmente. Norberto Bobbio, oltre alle cattedre che si conquistò, varie lauree *honoris causa*, in Italia e all'estero, per cui era un uomo titolatissimo. Poi il presidente Pertini lo nominò senatore a vita, ma lui, da intellettuale, sentiva il dovere di di entrare nel dibattito quotidiano, nel dibattito politico, sia pure da un profilo intellettuale. Ciò, evidentemente, comportava il non essere sempre amato o apprezzato da tutti. Come ha detto la senatrice D'Elia, che mi ha preceduto, era certamente un uomo di sinistra, che ha definito la sinistra in modo positivo. Il suo libro più venduto e più diffuso, «Destra e sinistra», una destra definita in negativo della sinistra. Io direi che era una sinistra, come secondo lui doveva essere e dovrebbe essere, e una destra come non dovrebbe essere e come, qualche volta, indubbiamente è stata. Da uomo di parte, però, indubbiamente ha anche scontentato la sua parte in tante circostanze: come quando fu attaccato dai pacifisti nel 1991,

con coraggio, affrontando appunto anche coloro che, pur della sua parte, lo attaccavano, mostrando appunto questo impegno civico verso l'ideale,

Comunico che, poiché non si è raggiunta l'unanimità nella Conferenza dei Capigruppo

Signor Presidente, Giulio Santagata, Ministro del secondo Governo Prodi, deputato della Repubblica dal 2001 al 2013, è stato un politico coraggioso e geniale ed è stato un uomo generoso e buono. È scomparso qualche giorno fa, il 5 gennaio, a Modena, città in cui ha vissuto, ha lavorato, dove ha cresciuto i suoi figli e che ha amato. Il suo nome resta legato alla più entusiasmante stagione del centrosinistra italiano e agli anni più fecondi del riformismo, prima con l'Ulivo, poi con l'Unione nel 2005: due campagne elettorali, due vittorie e, soprattutto, una grande speranza. Giulio è approdato alla politica in prima linea dopo essersi affermato nel suo lavoro di economista e, forse, anche per questo vi ha portato, con straordinaria vivacità, la voce e il punto di vista di quello che oggi chiamiamo la gente, il punto di vista dei cittadini e della società. D'altra parte, proprio questo è stato sempre il suo rovello: promuovere la partecipazione, fare in modo che della *res publica* tutti e tutte, in particolare i più giovani, abbiano voglia di interessarsi prendendovi parte. Lo ha fatto anche innovando fortemente le forme e le occasioni della partecipazione, per rendere vera la rappresentanza e produrre un consenso informato e consapevole. Nella sua veste di organizzatore delle campagne elettorali di Romano Prodi Giulio ha sostenuto e realizzato progetti straordinariamente innovativi, come la Fabbrica del programma e i Comitati per l'Italia che vogliamo. Entrambi strumenti di partecipazione paralleli alla vita e all'attività dei partiti e forse più attrattivi per chi è disponibile a un impegno più civico che direttamente politico e partitico. Parlare con le persone e ascoltarle, dando però loro certezza che una qualche vera disponibilità a recepire quello che dicono c'è. La partecipazione - diceva Giulio deve portare qualche risultato tangibile perché sia seria. Giulio si batteva, come hanno fatto gli ulivisti, per un riformismo radicale nelle idee, saldamente accompagnato dalla ricerca e dall'adozione di soluzioni praticabili e compatibili. Non si può più parlare solo alla pancia, ma non si può affidare ai tecnocrati la soluzione. Si devono tenere insieme le cose; dialogo, ascolto e competenza. poi l'altro suo rovello su cui è tornato di recente a parlare in un interessantissimo saggio pubblicato e presentato in questi mesi: la perdita la perdita di coesione sociale, che porta con sé la disuguaglianza che continua a crescere. La perdita di fiducia nella politica e nelle istituzioni; una piaga gravissima da combattere perché si sta bene solo se anche gli altri intorno a noi stanno bene. Giulio ha lavorato per costruire un Paese dove si sta bene a vivere e, citando le sue parole, sembra così facile da dire ed è così difficile da fare. Questa è la sfida che ci lancia ancora e che credo abbia molto da insegnare a chi ama la politica e a chi fa politica per amore del proprio Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, erano le 18,20 del 7 gennaio 1978 quando cinque militanti uscivano dalla sezione del Movimento sociale di Acca Larenzia per un volantinaggio. Nello stesso istante giungeva un gruppo armato sparando su di loro con armi automatiche. Tre persone cercarono rifugio dietro la porta blindata della sezione. Un ragazzo, Franco Bigonzetti, rimase ucciso sul colpo. Era iscritto al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia, non aveva che vent'anni. Morì, insieme ai suoi sogni di ventenne, vittima dell'odio cieco dei nuclei armati per il contropotere territoriale, organizzazione terroristica di estrema sinistra che rivendicò il *raid*. Francesco Ciavatta, studente diciottenne, ferito nell'agguato, tentò di fuggire, ma inseguito dagli aggressori fu colpito vilmente alla schiena e morì in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Alcuni mesi dopo il padre si uccise per la disperazione. Nelle ore che seguirono il vile agguato, un gruppo di attivisti organizzò un *sit-in* per le due giovani vite stroncate; stroncate dalla presunzione morale che chi ha idee differenti non ha diritto ad esprimerle e neanche a vivere. A loro si aggiunsero giornalisti, poliziotti, curiosi, gente comune. Probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta gettato nel sangue rappreso di una delle vittime, nacquero dei tafferugli, in seguito ai quali Stefano Recchioni, militante della sezione di Colle Oppio, fu colpito da un proiettile alla fronte e morì dopo due giorni di agonia. Le dinamiche e le responsabilità per la sua morte restano ancora irrisolte. Acca Larenzia è questo, colleghi. Acca Larenzia è sangue innocente versato per odio politico famiglie distrutte dal dolore della perdita di un figlio e dall'impossibilità, ancora oggi, di sapere chi sono stati gli assassini, il tutto in un silenzio delle istituzioni durato troppo a lungo. anni nessun tribunale ha trovato gli autori di quella strage, nessuna luce è stata fatta sulla mitraglietta Skorpion, una delle armi utilizzate nell'agguato, rinvenuta poi nel 1988 nel covo delle Brigate Rosse a Milano. Quella stessa arma fu utilizzata negli omicidi brigatisti dell'economista Ezio Tarantelli nel 1985, dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti nel 1986 e del senatore democristiano Roberto Ruffilli nel 1988. Di fronte a queste incognite, a queste domande e a questo dolore, davanti all'incubo di madri che sono morte dopo aver sperato inutilmente di conoscere il nome degli assassini dei loro figli, davanti all'indifferenza e all'odio ai quali quei morti sarebbero condannati, la risposta del Parlamento tutto dovrebbe essere solo la richiesta della verità. Oggi qui, insieme a Franco, Francesco e Stefano, voglio ricordare tutti quelli che hanno perso la vita in quel tempo tumultuoso, segnato dalla violenza politica e dalla discordia, perché la memoria ha un dovere imprescindibile e si parte dal ricordo, perché ricordare questa tragedia è un segno tangibile del nostro impegno per governare un sano processo di pacificazione nazionale, che ci porti a maturare una consapevolezza e un ricordo collettivo e condiviso in maniera trasversale. Abbiamo il dovere di imparare dagli orrori del passato e costruire un futuro in cui il dialogo e il rispetto reciproco prevalgano sulle divisioni ideologiche. Ho letto in queste ore i numerosi comunicati stampa da parte delle opposizioni, diversi articoli giornalistici in merito alle commemorazioni messe in atto domenica 7 gennaio: ricostruzioni fantasiose che parlano di saluti romani durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma capitale, alla presenza, fra l'altro, di rappresentanti delle istituzioni, come l'assessore alla cultura della Giunta capitolina, che ha espressamente negato la presenza di soggetti inneggianti con braccia tese. Ricostruzioni fantasiose, con attacchi a Fratelli d'Italia del tutto strumentali, perché si tratta di azioni compiute da persone non riconducibili né a Fratelli d'Italia, né al Governo. Allo stesso tempo, è fondamentale stigmatizzare coloro che ancora oggi adottano gesti simbolici legati agli estremismi del passato. Saluti romani e simboli simili non possono trovare spazio nella nostra società, come neanche la descrizione ossessiva e reale di chi vede saluti romani ovunque. Colleghi, vorremmo vedere lo stesso impegno nel chiedere che vengano finalmente individuati gli assassini di quella e di tutte le stragi degli anni di piombo. Non si può non apprendere la lezione di quel passato, che ha visto trionfare quell'odio che ha mietuto vittime innocenti, quell'odio che non va in alcun modo alimentato. Abbiamo il dovere di ricordare, chiedere ancora una volta verità e impegnarci perché mai più la politica sfoci nella violenza.

ed è morto il 5 gennaio nel carcere di Ancona. È stata una morte annunciata, per citare quel meraviglioso libro di Gabriel Garcia Marquez, perché Matteo Concetti aveva detto a tutti che che se fosse stato riportato in quella cella di isolamento si sarebbe suicidato e così è stato, poche ore dopo che la madre, che aveva tentato di percorrere ogni strada per togliere Matteo da quel luogo dove non doveva essere, aveva contattato anche la nostra collega Ilaria Cucchi, rivolgendosi alle istituzioni repubblicane e al Senato. Credo che dobbiamo ricordare Matteo Concetti in quest'Aula perché Matteo era, come alcune decine di migliaia di italiani, nelle mani della Repubblica e non è mai ammissibile che un nostro concittadino che è nelle mani della Repubblica esca da quelle mani morto. Quando questo accade, signora Presidente, è sempre un fallimento del nostro Paese ed è un fallimento ancor di più perché purtroppo le nostre carceri sono piene di persone come Matteo che non dovrebbero stare lì. lì. Matteo non era un criminale, non era un delinquente, era un ragazzo con una sindrome bipolare, che aveva fatto degli errori, che aveva avuto un'esperienza di tossicodipendenza, ma né la malattia psichiatrica, né la tossicodipendenza sono una buona ragione per essere nelle carceri dello Stato e tanti malati psichiatrici, tanti tossicodipendenti sono nelle nostre carceri perché purtroppo le nostre carceri sono diventate un ricettacolo di marginalità, di debolezza, perché semplicemente il nostro Stato, la nostra Repubblica di queste marginalità e di queste difficoltà non sa cos'altro fare. fare. Oggi ricordiamo la morte di un ragazzo che è morto per il semplice motivo che non doveva essere lì. Voglio dirlo anche al Governo e alla maggioranza, che utilizzano lo strumento carcerario in modo esagerato dall'inizio di questa legislatura; più volte abbiamo avuto l'occasione di dirlo in quest'Aula. Bisogna percorrere strade che svuotino le nostre carceri, che considerino la privazione della libertà personale un *extrema ratio* e non una soluzione ai problemi problemi sociali ai quali non riusciamo a fare fronte. Presenterò il mio atto di sindacato ispettivo, chiederò al ministro Nordio di spiegarmi perché quel ragazzo era lì, come sia possibile che un detenuto in isolamento abbia potuto impiccarsi, in che modo può averlo fatto se non avrebbe dovuto avere neanche i lacci delle scarpe, ma le dirò che qualsiasi cosa mi risponderà il Ministero della giustizia, come parlamentare di questo Paese che ai sensi della Costituzione rappresenta la Nazione, credo che con Matteo Concetti la Repubblica italiana abbia fallito.